intervengo per chiedere di avere quanto prima in Aula il signor ministro Antonio Di Pietro: quanto è successo ieri sera durante la trasmissione «Porta a Porta» è stato infatti offensivo e umiliante sia per il Governo, sia per questo Parlamento. Il ministro Di Pietro non è stato all'altezza del ruolo che riveste, ha detto che era favorevole ad un Governo con un numero massimo di 15 Ministri, ma mi sembra che sieda in un Consiglio dei ministri ben più numeroso; ha detto che è contrario al finanziamento elettorale dei partiti, finanziamento che non mi risulta la sua lista abbia mai rifiutato; ha detto che è sbagliato percepire il rimborso delle spese di viaggio perché come Ministro ha già tutto pagato, ma anche a queste non ha mai rinunciato. Non è dignitoso per un Ministro accedere e scendere ad un livello così basso e con tanta leggerezza. Vorrei ringraziare, invece, colleghi, il giornalista presente a quella trasmissione, perché è stato l'unico che ha dimostrato buonsenso e in maniera convinta ha difeso la dignità delle istituzioni e la verità delle cose.

Sud. Non mi sento però di tacere e, visto che non lo ha fatto nessuno, gli esprimo la mia solidarietà per l'attacco che ha subito l'altra sera durante la trasmissione «Ballarò» e, pur appartenendo all'opposizione, lamento che nessuno in quest'Aula si sia alzato a dare questo segno di dignità rispetto ad un collega messo nel mirino.

a Roma, dopo i tragici eventi che lo hanno colpito in Afghanistan. Nessun esponente del Governo, nessun esponente della maggioranza e della minoranza ha accolto, se delegato, il giovane uomo,

Neanche il Presidente della Repubblica, che arrivava in quel momento, è stato avvertito che era concomitante l'arrivo del giovane militare. Credo che questo segnale sia veramente vergognoso

Presidente, mi scusi, ma quest'Aula non credo si possa sottrarre dal manifestare solidarietà anche al suo Presidente, perché quanto oggi è pubblicato a pagina 12 del giornale «la Repubblica» ha davvero bisogno di essere stigmatizzato: non si può pubblicare la foto del nostro Presidente in missione ufficiale in Canada dicendo che ha caricato sull'aereo blu sull'aereo blu suo cugino. È un fatto davvero disdicevole. La politica oggi è attraversata da un momento di grande difficoltà, probabilmente anche perché la modifica della forma dello Stato è stata rinviata da un voto referendario che non ha apprezzato gli sforzi che nella precedente legislatura erano stati fatti. È un problema che si riversa sulla responsabilità del Parlamento e del Capo dello Stato, che oggi probabilmente farebbe bene ricercando altri precedenti, come ci furono nel 1994 - a sciogliere il Parlamento e a far sì, come ha detto il ministro Di Pietro stamattina in Parlamento, che vi sia una maggioranza più coesa, quale che sia, che possa affrontare il problema della riforma dello Stato e della modifica della forma di Governo, così da non consentire che le istituzioni, prima fra tutte il nostro Presidente, siano dileggiate da un giornale della Nazione. Un giornale che, come altri, si sta segnalando all'opinione pubblica

La ringrazio di cuore, senatore. Debbo dire che, una volta tanto, quantomeno la verità, la risposta, c'è in quel giornale. Apprezzo quello che ha detto, ma direi che rispetto a questi interventi

Il Governo, come preannunciato nella seduta pomeridiana di ieri, ha presentato ieri sera stessa un nuovo emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato. L'emendamento è già stato stampato e distribuito. Come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, eventuali subemendamenti - c'è un punto solo su quell'emendamento - potranno essere presentati entro le ore 10,30. Nell'interesse della discussione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, la Presidenza ha rinviato alla 5a Commissione permanente l'articolo 1 del disegno di legge e il nuovo emendamento ad esso riferito. La Commissione bilancio, che è autorizzata a convocarsi immediatamente, riferirà all'Assemblea alle ore 11. Nel frattempo l'Assemblea riprenderà la discussione del disegno di legge n. 1532, concernente lo sportello unico delle imprese.

È un modo sintetico di dirlo. La sospensione non può essere concessa con una motivazione della quale ancora non sono conosciute le connotazioni, come l'eventuale presentazione di un emendamento,

a dire 2.000 miliardi di vecchie lire. Non si tratta di una lieve modifica, di una correzione di rubrica. Non solo: all'emendamento sono allegate dieci pagine di relazione tecnica.

con un tempo non sufficiente, ma con una seduta che abbia tutta la sua regolarità, i suoi crismi e la possibilità di espletarsi e di evolversi. Ragion per cui, signor Presidente, la mia proposta è di rinviare in Commissione

fare le cose di fretta, perché non si consente al Parlamento di verificare e tutelare il diritto dei cittadini in ordine ai documenti di contabilità. Il Governo farebbe bene a non fare sedute notturne, al buio e negli anfratti dei Ministeri, ma a venire in Parlamento a rendere noti

e l'orientamento, anzi l'invito dell'Aula ieri sera, al di fuori delle divisioni politiche, era quello di andare in Commissione.

Presidente, condivido la sua proposta relativamente ai tempi assegnati alla Commissione bilancio. Tuttavia volevo farle presente che la sua proposta di riprendere

rimasti aperti. Invece di una sospensione di mezz'ora, nel caso non intendesse accogliere la proposta del senatore Ripamonti,

lei stia ipotizzando un percorso improponibile. Non vogliamo fare commenti sul fatto che non si riescono a gestire i lavori dell'Aula, certo non per colpa della Presidenza o dei funzionari, ma indubbiamente perché la maggioranza è in ordine sparso sui temi che si devono affrontare. Lo abbiamo colto anche nel brevissimo dibattito di questa mattina: c'è chi vorrebbe andare avanti e chi non vorrebbe, c'è chi è d'accordo per l'avvio dello sportello unico, chi è contrario chi non vuole che si vada avanti perché, se la Commissione bilancio - e mi sembra anche molto correttamente - deve lavorare, i suoi membri non possono partecipare ai lavori d'Aula. Quando si arriva a questi ingorghi è inutile muoversi più di tanto, perché si rischia di complicare ancora di più la situazione. Se c'è bisogno di tempo, si dia questo tempo, si sospenda l'Assemblea, si riprendano serenamente i lavori, onde evitare, signor Presidente (e glielo dico con il senso di rispetto e di orgoglio che ho nei confronti dell'Assemblea

nel modo migliore, cioè in maniera collaborativa e nel rispetto dei lavori di quest'Aula parlamentare. Signor Presidente, quello che avevamo già annunciato ieri si è materializzato con la presentazione dell'emendamento del Governo. Crediamo che per un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari sia opportuno consentire

lo stato di previsione delle entrate e la Tabella 2. Si tratta di fare una valutazione su tutta la politica dell'entrata, in questo caso sulle entrate che derivano dall'imposta sulle società. Occorre, quindi, consentire alla Commissione bilancio di fare le proprie, adeguate valutazioni, determinando le condizioni affinché l'Assemblea possa serenamente affrontare il provvedimento la prossima settimana. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione bilancio esaminasse l'emendamento nella mattinata odierna, con tutta serenità, e che

molto brevemente solo per chiedere che lei e i Gruppi, fatte salve le esigenze che sono state manifestate, teniate conto della necessità che il Governo possa effettivamente riferire sulla situazione in Birmania, come programmato, e che si consideri ciò nell'organizzare il complesso dei lavori. innanzitutto dal punto di vista procedurale e poi da quello politico. Dal punto di vista procedurale, Presidente, se lei decide - come è stato segnalato anche dai Verdi - di continuare nei lavori parlamentari, è evidente che, essendo riunita la Commissione bilancio,

questione difficilmente è emendabile in tempi brevi, anche perché occorre una relazione tecnica e quant'altro. Tecnicamente, in un'ora e mezza non è possibile. La Ragioneria dello Stato

dopo un percorso politico e procedurale quanto meno discutibile. Se lei forza la mano, è evidente che dovrà registrare una reazione da parte dell'opposizione.

di buona sostanza, nel senso della quantificazione, ha necessità di essere profondamente discusso. È chiaro, infatti, che esso va a variare il saldo netto da finanziare. Occorre vedere se detta variazione ha

Signor Presidente, la Commissione bilancio ha concluso pochi minuti fa i suoi lavori. Vi è stato un dibattito approfondito sull'emendamento 1.Tab.1.600, presentato ieri sera dal Governo, e si è pervenuti a un voto favorevole sull'emendamento stesso. la maggioranza ha ritenuto di doversi esprimere favorevolmente, poiché nel momento in cui il Governo, come ieri sera ha preannunziato in quest'Aula, è venuto a conoscenza del dato delle maggiori entrate IRES, pari a 900 milioni di euro, sarebbe stato strano e incomprensibile non aggiornare il dato stesso, che era già stato oggetto di un emendamento

alla correttezza e all'esaustività di informazioni riguardanti il minor gettito rilevato sull'IRE e anche alcune voci di riduzione di spesa, in particolare per quanto riguarda le risorse proprie, il contributo cioè che

Vi sono alcuni elementi che devono essere necessariamente approfonditi per valutare, ad esempio, quanta parte di questo maggiore gettito, molto rilevante, complessivamente registrato con l'assestamento sia di carattere strutturale e quanta invece sia legata a fattori contingenti. La conclusione alla quale mi sembra siamo pervenuti, sui cui si è registrata una condivisione generalizzata, è che esiste lo strumento attraverso il quale operare tali approfondimenti e mettere il Parlamento nelle condizioni di valutare la destinazione di questo extragettito, anche relativamente agli strumenti della manovra finanziaria che saranno varati nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri. Questo strumento è costituito dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria dell'anno scorso, che, oltre a indicare in modo preciso la destinazione dell'eventuale extragettito che fosse stato rilevato, indica con precisione che entro il 30 settembre, quindi siamo in tempo, il Ministro dell'economia presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione (e poi, nel complesso dell'esame della norma, si evince che non si riferisce ovviamente solo ai ai risultati della lotta all'evasione) quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzione della pressione fiscale, ai sensi del comma 4. Ricordo appunto che questo comma fa riferimento alla finalizzazione relativamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di equità sociale, dando priorità a misure di sostegno al reddito di soggetti incapienti, ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse. quindi che questa obiezione possa essere superata attraverso questa sollecitazione, che mi auguro il Governo faccia propria, consistente appunto nella necessità di presentare, unitamente mi auguro ai provvedimenti della manovra di bilancio, questa relazione al Parlamento, in tal modo permettendoci di fare valutazioni coerenti appunto con la legislazione vigente. Poi sono state sollevate altre obiezioni relative a un supposto intendimento del Governo di predisporre la copertura per il decreto di cui si parla e sulla sulla legittimità della utilizzabilità di queste maggiori entrate e minori spese, quindi di queste maggiori disponibilità per coprire provvedimenti che eventualmente il Governo si determinasse ad adottare, ma di tale argomento parleremo nella sede propria, quella appunto dell'esame degli eventuali provvedimenti che saranno adottati, e non mi sembra che in questa fase di esame dell'assestamento si possa fare un processo alle intenzioni. Lo vedremo quando sarà

convertito in legge i primi d'agosto. Vedremo se nei prossimi giorni il Governo presenterà un decreto come quello che viene ipotizzato e discuteremo

Presidente, esprime un parere contrario sull'ordine del giorno G1, in quanto non può assolutamente ritenere che ci sia stata alcuna violazione delle norme e delle prassi di corretta amministrazione per quel che riguarda la contabilità pubblica.

delle rendite finanziarie. Se il Parlamento intende assumere un atto d'indirizzo, può farlo oggi confermando ciò che hanno sostenuto il presidente Prodi e il Ministro dell'economia,

decisione che andava in senso assolutamente contrario rispetto a quanto sostenuto oggi dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia. Se il Senato intende supportare la proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia, può farlo accogliendo un ordine del giorno che smentisce ciò che è stato approvato in occasione della discussione del DPEF.

L'emendamento approvato in Commissione che oggi voteremo in Aula porta ad una grossa modificazione degli stanziamenti per i vari Ministeri. In particolare, vi è una grossa riduzione ‑ stiamo parlando del 2007

Adesso vorrei capire dal relatore cosa c'entrano le decisioni che andremo ad assumere rispetto all'attualità di una riduzione degli stati di previsione per il Ministero della difesa e della necessità di garantire queste risorse oggi e non con la prossima finanziaria.

ma ritengo, per le ragioni che ho esposto in sede di discussione generale, che sia stata modificata la cornice della legge di assestamento, vi è una grave violazione, vi è anche una sanatoria, come abbiamo visto, nel rendiconto rispetto alle autorizzazioni. Ritengo che le argomentazioni che ha portato il relatore Legnini non siano sufficienti, perché non basta dire che il Governo era impegnato dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria, quando sappiamo bene che questo gettito non deriva da lotta all'evasione. Infatti stiamo parlando di imposta sulle società, quindi questo è stato determinato da interventi legislativi: non c'è nessuna lotta all'evasione, non confondiamo le idee agli italiani.

il parere contrario sugli stessi. Ribadisco il fatto che il primo ordine del giorno, il G1 (testo 2), si riferisce appunto ad una previsione di utilizzo ad una previsione di utilizzo di queste maggiori risorse nel contesto della manovra di finanza pubblica che è in via di predisposizione e quindi tende ad anticipare una discussione che sarà fatta Il secondo e il terzo ordine del giorno si riferiscono al contenuto della manovra finanziaria prossima ventura di cui si sta discutendo in questi giorni e per la stessa ragione ho ritenuto e ritengo che sia inopportuno che oggi il Senato venga

solo formale, ma anche politica, in questo momento di discussione della politica economica e della presentazione del disegno di

premesso che: il Governo ha presentato un emendamento approvato in Commissione, che determina variazioni degli stati di previsione e in particolare una riduzione dello stato di previsione del Ministro della difesa, in più occasioni i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali sono stato oggetti di aggressioni che hanno portato, purtroppo, a feriti anche gravi, impegna il Governo: a confermare comunque gli impegni assunti nelle missioni internazionali per la costruzione della pace e della stabilità e a garantire le risorse per i supporti logistici e tecnologici nonché per gli armamenti necessari a garantire la sicurezza di tutti coloro che operano nel contesto di tali missioni». Si chiede che il Governo confermi quanto è stato deciso. Sicuramente in questo emendamento vi è una pesante riduzione degli stanziamenti; se queste riduzioni dovessero andare ad incidere sulla sicurezza dei nostri militari,

Presidente, l'emendamento presentato dal Governo nel corso della discussione dell'assestamento presenta delle variazioni di un certo rilievo, anche se modeste e contenute rispetto alle altre variazioni relative al saldo netto da finanziare operate aumento delle entrate registrato negli ultimi mesi e previsto per l'anno in corso: si tratta di aggiustamenti rispetto ai capitoli, e quindi all'unità previsionale di base, del Ministero della difesa. Non è dato di capire perché l'emendamento faccia riferimento a quella formalità e a quella scarsa possibilità di lettura

della rappresentanza politica nazionale, dai giornali, per quella presenza qualificatissima (un po' oggetto di confronto per quel che riguarda

una specifica indicazione in proposito. È un ordine del giorno di estrema prudenza, pure necessaria, che si

colleghi della maggioranza non ci conforteranno con una loro opinione in proposito mi fa ben capire come c'è, sul tema delle risorse per il comparto della Difesa, un'attenzione soltanto in certi momenti e una sconfortante disattenzione in momenti come questo. Ma si sa, la vita politica è fatta di frangenti in cui è molto più importante pensare che la seduta possa andare a finire tra mezz'ora, che non andare a discutere su come utilizzare risorse che sappiamo essere sostanziose, come evidenziato dagli emendamenti presentati dal Governo. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo dopo.

l'ordine del giorno G2, testé letto in Aula dal senatore Calderoli, risponde ad intenti lodevoli che credo non si possano disconoscere, salvo il fatto che forse sottintende una preoccupazione che non è giustificata dalle premesse. Non ho in questo momento in mano i dati analitici dell'assestamento di bilancio esposti dal Ministero della difesa, ma credo che in sostanza essi quasi si compensino o, se o, se vogliamo essere più precisi, determinino a saldo una riduzione dello stato di previsione dell'ordine di 3 milioni di euro, ossia di una portata evidentemente molto modesta. D'altra parte, questi spostamenti di bilancio non riguardano le missioni internazionali, che - come tutti sappiamo, per l'ampiezza che è stata data in quest'Aula ai provvedimenti legislativi in proposito - vengono finanziate ora in ragione annuale con atti legislativi specifici. Credo, quindi, che forse il senatore Calderoli potrebbe non insistere nella richiesta di votazione, ma se questo sommesso invito non avesse successo voterò contro l'ordine del giorno, appunto perché esprime nel dispositivo una preoccupazione che non è giustificata dalle premesse che dovrebbero motivarla. Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno G2 anche per aver ascoltato le espressioni, ancorché garbate, del senatore Zanone. Vorrei capire dal Governo se l'ordine del giorno viene letto dalla firma o viene letto nel contenuto. In apertura dei lavori di oggi il senatore Giulio Marini, appartenente al Gruppo Forza Italia, ha sollevato una questione riguardante il comportamento delle istituzioni della Repubblica nei confronti di un soldato ferito in Afghanistan, che è tornato a Roma e non ha trovato uno straccio di carica istituzionale ad accoglierlo. Credo che abbia fatto bene il collega Marini a denunciare e farebbe malissimo il Senato della Repubblica a non rappresentare al Governo che si è trattato di un fatto grave. Ora, il Governo, per metterci qualcosa di suo in termini negativi, dice no

che il Governo si impegni a mantenere propri impegni. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo qual è il delitto che si commette contro la democrazia nel pretendere che il Governo mantenga la propria parola, perché delle due l'una:

di persuasione morale nei confronti del Governo, perché davvero dire no a quest'ordine del giorno significa contraddire tutto quello che sta dicendo l'Esecutivo in tema di politica estera. Posso capire che sono questioni che incidono anche sulla coesione della maggioranza, ma non si è mai visto un Governo che dice no a se stesso.

Vi si chiede di fare una cosa che dite che state già facendo, per cui non capisco quale sia la difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno G2. Non è piuttosto il modo di destare il sospetto che non avete davvero intenzione di farla? Tre milioni di euro, senatore Zanone, sono una piccola cifra, ma la politica è fatta anche di segnali. In un momento in cui i nostri soldati all'estero, in modo particolare in Afghanistan, sono particolarmente esposti perché si sviluppa un'offensiva dei talebani che investe le aree da essi presidiate; nel momento in cui la pressione della missione ISAF induce i talebani a sgombrare i territori dove finora erano fortemente trincerati per cercare scampo in aree fino a ieri meno investite dalla loro attività e che sono presidiate da soldati italiani; in un momento in cui l'opinione pubblica è giustamente allarmata per il recente episodio che ha portato al ferimento grave di uno dei nostri soldati e a quello più lieve di un altro, qual è il segnale simbolico che mandiamo? Quello della riduzione degli stanziamenti per la difesa? Né vale, senatore Zanone, il dire il nostro impegno in Afghanistan è finanziato con altro separato provvedimento. Chiedo al Governo: questo altro separato provvedimento concerne le spese di funzionamento della nostra missione in Afghanistan o riguarda anche l'attrezzatura generale, l'addestramento, le dotazioni logistiche, l'armamento, il rinnovamento dei mezzi, che sono ciò che sta prima del momento in cui i soldati partono per l'Afghanistan, ma che incide in modo decisivo sulle condizioni di sicurezza nelle quali essi si trovano ad operare? I giubbotti antiproiettile li compriamo con le dotazioni specifiche per l'Afghanistan o con le dotazioni generali del Ministero della difesa? I carri armati, gli elicotteri, li compriamo con le dotazioni per l'Afghanistan o con quelle del Ministero della difesa? In un momento in cui il ministro Parisi afferma di non avere la benzina per far compiere l'addestramento ai soldati (e voi sapete che la prima difesa del soldato è l'allenamento fisico e l'addestramento specifico); in un momento in cui non siamo in grado di garantire condizioni ottimali di addestramento specifico e di allenamento fisico ai nostri soldati; in un momento in cui il che l'usura dei mezzi è tale da richiedere la sostituzione di quelli inviati in Afghanistan (perché un anno in Afghanistan comporta un'usura pari a dieci anni di utilizzo del mezzo in Italia); in un momento in cui ci dice che senza 600 milioni di euro di nuovi stanziamenti addizionali è pronto a chiudere il Ministero della difesa e a buttare le chiavi nel Tevere; in un momento così, il segnale che lanciamo ai nostri soldati, all'opinione pubblica e al Paese è un segnale distruttivo. Vorrei invitare il Governo a ripensare il parere che ha dato.

qualsiasi partito usa espressioni di grande solidarietà nei confronti dei nostri soldati che svolgono operazioni di pace, facendo un distinguo fra l'aspetto politico - alcuni - e l'aspetto realizzatore che è costituito dall'opera dei nostri uomini. Chiunque ne fa gli elogi, chiunque afferma che dobbiamo essere solidali con loro e chiunque dice che debbono essere adeguatamente equipaggiati. Quando poi capita un incidente, il clamore è fortissimo: evviva i nostri soldati; il nostro cuore è vicino ai nostri soldati; i nostri soldati vanno sostenuti; va elogiato il loro impegno che dà tanto prestigio - questa volta sul serio - al nostro Paese; anzi, forse l'unico biglietto da visita che dà veramente prestigio al Paese è proprio l'operato di questi nostri uomini.

proteggendo ed equipaggiando adeguatamente i nostri uomini, se è vero che siete così solerti nel preoccuparvi del sostegno *bipartisan* nei loro confronti. Dice anche di incentrare lo sforzo nell'acquisizione di mezzi e di strumenti che possano facilitarne la protezione oppure l'altra attività da tutti auspicata, cioè la prevenzione dell'attacco, in modo da evitare che la reazione venga a volte considerata esagerata, spropositata o altre facezie del genere.

il logorio di un mezzo di protezione o di movimento o di difesa in un anno in Afghanistan è pari al logorio di dieci anni degli stessi mezzi in Italia, e a un certo punto - come ha ricordato il minacciato di chiudere il Ministero perché non è possibile continuare in quel modo; e così fa il suo Sottosegretario. Ebbene, nel momento in cui il componente responsabile della difesa del Governo fa un chiaro appello *urbi et orbi* perché si consideri con serietà questo impegno, il Sottosegretario all'economia è contrario e anche altri che hanno parlato dicono che le operazioni di pace vengono finanziate specificatamente e che non hanno niente a che vedere con un finanziamento generalizzato di indurimento della protezione, sbagliando, perché se ieri era presente al discorso del Ministro avrà sentito proprio dire che i 1.000 miliardi di copertura delle spese per le operazioni di pace servono soltanto per le spese vive, ma non riguardano la protezione e gli equipaggiamenti. equipaggiamenti. Nonostante tutti chiacchieriate, perché nel momento in cui dovete esprimere solidarietà ai soldati allora fate la faccia seria e compunta, nel momento in cui si parla di aiutarli concretamente continuate a chiacchierare dando un bell'esempio di serietà, vi chiedo: è possibile che il Governo dica una volta una cosa e poi ne dica un'altra? È possibile che la maggioranza esprima il desiderio autentico e serio di proteggere e sostenere i nostri uomini e poi, nel momento in cui si tratta di dare quattro soldi

potrà essere speso meglio di quello che spenderemo per proteggere i nostri soldati ai quali tutti esprimono grande solidarietà e grande stima.

all'ordine del giorno G2 presentato dal collega Calderoli. Si tratta, infatti, di un ordine del giorno a mio modo di vedere estremamente condivisibile, perché - come hanno riferito e sottolineato alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto gli impegni dei nostri militari, che si svolgono nelle zone più difficili e più impegnative, devono trovare una grande consistenza e un grande supporto.

in situazioni e in aree del mondo particolarmente tribolate. Direi che da questo punto di vista vi è un consenso, vi è una partecipazione, è un coinvolgimento estremamente puntuale per quello che i nostri militari sono in grado di svolgere Mi è capitato di visitare i luoghi dove i nostri militari svolgono queste missioni e ho sempre potuto constatare non solo il grande impegno, la grande professionalità, la grande dedizione

proprio perché il mandato che loro hanno ricevuto dal Parlamento è collegato all'impegno per la pace,

che condividiamo e che abbiamo avuto la possibilità di vedere e di verificare, credo allora che ciò che è contenuto nel dispositivo dell'ordine del giorno del senatore Calderoli sia una doverosa conferma di quello che noi dobbiamo assumere e di quello che il Governo deve impegnarsi a fare nei confronti dell'attività che i nostri militari svolgono nelle missioni internazionali. Come è scritto nel dispositivo, si tratta di «missioni internazionali per la costruzione della pace e della stabilità». Dobbiamo allora garantire tutti gli strumenti, tutte le modalità, tutte le circostanze necessarie per consentire uno svolgimento adeguato, efficace efficace e costruttivo di queste nostre missioni e di questi nostri impegni con i nostri militari. È necessario fornire le risorse - come è scritto nell'ordine del giorno per i supporti logistici, per tutte le tecnologie, per gli armamenti necessari, nonché (e questo è un elemento veramente fondamentale che voglio sottolineare) per garantire la sicurezza che deve essere tale per tutti coloro che operano appunto in quel contesto. La sicurezza è un elemento fondamentale. Dobbiamo fare in modo che siano a disposizione: lo abbiamo anche evidenziato in altre circostanze, in altri momenti. Abbiamo supportato in modo particolare particolare l'esigenza di fornire tutte le attrezzature tecnologicamente più avanzate e più adeguate per consentire le capacità operative dei nostri militari

Sarebbe una cosa assolutamente disdicevole e non comprensibile se il Governo non potesse o non dovesse accettare non potesse o non dovesse accettare questo ordine del giorno, perché verrebbe meno qualcosa di fondamentalmente elementare

si avvicina agli stessi banchi).* Senatore Legnini, lei non è autorizzato a fare che il relatore, non può fare il segretario o il Presidente: non c'è il cumulo delle cariche.

credo sarebbe più utile, anche dal punto di vista formale, se lei volgesse lo sguardo a centottanta gradi e non soltanto da una parte.

relazione al secondo punto del dispositivo il Senato non può tornare ad assumere decisioni sulle quali si è già espresso. Accogliendo questa osservazione, sono disponibile a rinunciare al secondo punto del dispositivo limitandomi ad impegnare il Governo «a ribadire le volontà espresse in premessa», ovvero quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia rispetto alla manovra

non modifico il mio parere, che resta contrario per le ragioni che ho ampiamente esposto, ovvero che sul punto vi è una deliberazione di questa Assemblea

*(LNP)*. Signor Presidente, a questo punto devo ritenere che il Sottosegretario non concordi e non attribuisca fiducia al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia. Ma quello che è ancora più certo è che quanto è stato dichiarato (stiamo parlando di un ordine del giorno, non di un articolo), vale a dire che non si sarebbe

il buonsenso per il timore che la maggioranza possa dividersi e qualcuno possa dire di no e far emergere che sono di più quelli che vogliono aumentarle le tasse, altro che restituirle ai nostri cittadini! *(Applausi dai Gruppi

il Senato della Repubblica nella sede propria, la risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, tuttora valida, ha espresso un indirizzo molto preciso e molto chiaro. In tema di pressione fiscale

un termine di indirizzo generale. sempre nella stessa risoluzione la maggioranza ha detto che se ci sono nuove spese da fare, e ci saranno naturalmente, esse devono essere finanziate attraverso corrispondenti risparmi di spesa.

sulle rendite da capitale agiscono due aliquote di prelievo, una del 27 per cento sui conti correnti della povera gente ed una del 12,5, per esempio sulle *stock option* dei grandi *manager* - la risoluzione

per esempio, a favore dei redditi medio-bassi con una riduzione dell'IRPEF o a favore delle imprese con una riduzione dell'IRAP e così via. Il Governo sceglierà, ma gli indirizzi su questo punto sono già stati formulati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Trovo assurdo che adesso il Senato frettolosamente su un ordine del giorno di tipo chiaramente strumentale

all'attenzione dell'Assemblea il problema delle cosiddette rendite finanziarie, collegato all'aumento della pressione fiscale. È innegabile che la pressione fiscale sia aumentata del 2,5 ed è innegabile che è stata sbagliata la manovra di finanza pubblica dello scorso anno. Ciò ha determinato un eccesso di pressione fiscale che la maggioranza non riesce più ad arrestare. Una parte della maggioranza ha posto un vincolo, in particolare lo ha fatto il senatore Dini, chiedendo di non intervenire sulle tassazioni delle rendite, facendo una proposta di buon senso. È il momento sbagliato per intervenire sulle rendite finanziarie ove lo si volesse fare perché le decisioni assunte nel mese di luglio sono state travolte da quanto è successo nei mesi successivi; stiamo ancora aspettando la Nota di variazione che dovrà essere presentata dallo stesso Governo per aggiustare le previsioni sbagliate; è intervenuta la crisi dei mercati finanziari con la questione dei mutui *subprime*. Tutti questi elementi devono essere tenuti in considerazione. Allora, la questione centrale, posta dal senatore Calderoli, è un aumento eccessivo della pressione fiscale insieme ad una misura, come quella dell'intervento sulle rendite finanziarie, che travolgerebbe la questione dei

favorendo naturalmente un modesto *capital gain* piuttosto che una tassazione al 20 per cento. Questo è il rischio che voi ponete all'industria del risparmio italiano. Questa misura andrebbe collegata ad una tassazione degli affitti con una cedolare secca, sulla quale avete fatto tante promesse e nessun intervento serio. Per queste ragioni ritengo che l'ordine del giorno G3 del senatore Calderoli debba essere

tassare in modo diverso il circolante rispetto alle nuove emissioni, è come se tassassimo i salami prodotti da oggi in avanti con un'aliquota IVA diversa da quelli vecchi. Non è possibile, il prodotto è lo stesso. Il risultato netto è che aumenterebbe la tassazione, con un prelievo fiscale a danno sì dei grandi risparmiatori, ma soprattutto dei piccoli, degli impiegati, degli operai e dei pensionati, categorie che detengono risparmio, anche se la sinistra a volte si dimentica che esistono come categoria e come risparmiatori. Detto questo, sarebbe assolutamente improvvido: per gli effetti economici sui cittadini avrebbe un significato di maggiore pressione fiscale. Sarebbe sbagliato nell'attuale situazione economica, in quanto viviamo in un momento nel quale occorre incentivare il risparmio e non scoraggiarlo, anche con riferimento agli investimenti esteri. Abbiamo un PIL in diminuzione ed un aumento delle rendite, soprattutto preannunciato, significa far scappare gli investitori e pregiudicare le possibilità di sviluppo del Paese. Il fatto che si riproponga oggi il problema con questo ordine del giorno manifesta il senso della sua urgenza,

che la maggioranza aveva avanzato anche la proposta di vendere l'oro della Banca d'Italia, proposta sulla quale il Governo è rimasto negativamente e colpevolmente in silenzio.

comunico che la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, del in materia di sicurezza stradale, in scadenza mercoledì 3 ottobre.

il senatore Dini, che mi sembrava molto interessato alla materia. Dalla stampa si apprende che si sarebbe raggiunto un patto perché il Presidente del Consiglio non aumenti le

i drammatici sviluppi della situazione in Myanmar destano nel Governo italiano la più viva preoccupazione. Voglio però preliminarmente ripercorrere, seppure in maniera sintetica, i passaggi salienti dei 40 giorni di proteste popolari contro la giunta militare di Myanmar che hanno portato agli eventi delle ultime ore. Il 15 agosto è raddoppiato, senza preavviso, il prezzo del diesel e quintuplicato quello del gas naturale con la paralisi del trasporto pubblico nell'ex capitale Yangon. Il 23 agosto sono stati arrestati 13 dissidenti che rischiano fino a 20 anni di carcere; il 28 agosto, dopo due settimane di proteste organizzate da attivisti e da gruppi di opposizione al regime, per la prima volta, si uniscono alle manifestazioni anche i monaci buddisti; il 5 settembre, militari sparano colpi di avvertimento per fermare 500 monaci che manifestavano a Pakokku, a 600 chilometri a nord-ovest di Yangon. Il 6 settembre diverse centinaia di monaci tengono in ostaggio quattro funzionari governativi e bruciano la loro auto; l'11 settembre i monaci minacciano di continuare la protesta fino a quando la giunta non chiederà scusa per l'intervento di Pakokku; il 16 settembre sono arrestati a Sittwe due monaci; il 23 settembre i monaci in corteo sostano davanti alla casa del premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, che è agli arresti domiciliari e che si mostra in quella occasione in pubblico. Il 20 settembre, dopo tre giorni di barricate, a circa 500 monaci è permesso di entrare a pregare nella pagoda di Shwedagon, a Yangon, il luogo dove sono custodite le reliquie più sacre del Myanmar. Il 23 settembre anche monache buddiste aderiscono per la prima volta alla protesta dei confratelli nella pagoda di Shwedagon; il 24 settembre in 100.000 manifestano nell'*ex* capitale e questa è la più grande dimostrazione dal 1988, quando la giunta militare prende il potere stroncando nel sangue una rivolta studentesca. Mentre sino a qualche giorno fa le autorità birmane avevano preferito mantenere un controllo a distanza delle proteste limitandosi a filmare i cortei e a compiere arresti sporadici di dimostranti, negli ultimi 3-4 giorni l'ampliarsi della protesta popolare, dopo l'introduzione del coprifuoco, ha portato ad una degenerazione violenta delle repressioni, benché il movimento popolare stesso fosse dichiaratamente ispirato ad una sostanziale adesione - anche per volere degli stessi monaci - ai princìpi della non violenza. L'Italia ha adottato, fin dal mese di settembre, un atteggiamento di coerente rigore di fronte a questi eventi. In sede bilaterale, già all'inizio di settembre siamo stati tra i primi Paesi dell'Unione Europea ad effettuare un passo formale con l'ambasciata di Myanmar a Roma. Un passo in cui si era manifestato, anche sulla base di quanto comunicato da parte dei capi missione dell'Unione Europea residenti in Yangon, del rammarico e della preoccupazione per il sostanziale fallimento della Convenzione nazionale in Myanmar nata con l'obiettivo di dare avvio ad un reale processo di riconciliazione nazionale e di apertura democratica nel Paese. Al tempo stesso, avevamo espresso la nostra condanna per le repressioni allora attuate dalla giunta militare al potere, deplorato gli arresti di cittadini birmani avvenuti nel corso delle dimostrazioni pacifiche pacifiche e stigmatizzato la perdurante detenzione del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, così come di altri dirigenti dell'opposizione e di prigionieri politici. Il 25 settembre scorso il competente Sottosegretario agli affari esteri ha convocato alla Farnesina l'incaricato d'affari dell'ambasciata di Myanmar a Roma, titolare della stessa rappresentanza diplomatica in assenza dell'ambasciatore, al quale a nome del Governo ha chiesto di trasmettere alla giunta militare al potere in Birmania la richiesta del Governo italiano di aprire un dialogo immediato con i monaci, con i membri della *National League for Democracy* e con tutta l'opposizione birmana e di non far corso ad alcuna forma di violenza nei confronti delle dimostrazioni pacifiche e non violente di questi giorni. Il Sottosegretario ha inoltre stigmatizzato gli episodi di repressione che hanno portato all'arresto di decine di manifestanti ed alle condanne arbitrarie di numerosi sindacalisti ed oppositori del regime, reiterando la richiesta di libertà immediata al premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi anni segregata agli arresti domiciliari, insieme a quella del rilascio di prigionieri politici detenuti in modo arbitrario. All'incaricato d'affari birmano è stato anche fatto presente che il Senato della Repubblica il 13 settembre scorso ha approvato una mozione che impegna il Governo italiano ad adoperarsi a questo fine, nonché ad operare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla posizione comune dell'Unione Europea e per richiamare le autorità governative birmane al rispetto dei diritti umani. Alla luce degli ultimi sviluppi, abbiamo poi deciso di sospendere la partecipazione di due diplomatici birmani ad un corso di formazione in materia di *institution building* destinato a Paesi della regione che si terrà il mese di ottobre in Italia. II presidente del Consiglio Prodi e il ministro degli affari esteri D'Alema, a New York per l'Assemblea generale dell'ONU, hanno espresso ripetutamente, nei giorni scorsi, la solidarietà del nostro Paese con le manifestazioni per la democrazia in corso a Myanmar, e chiesto alla giunta militare di rispettare il diritto del suo popolo di esprimersi e di protestare. Da ultimo, nella giornata di ieri, hanno esplicitamente ribadito come il nostro Paese si impegnerà in tutti i fori multilaterali e all'interno dell'Unione Europea affinché le violazioni dei diritti umani in atto in Myanmar cessino immediatamente. In questo spirito, il nostro Paese sta operando per promuovere, in tutti gli ambiti opportuni, dalle Nazioni Unite all'Unione Europea, tutte le iniziative necessarie per sostenere il desiderio di libertà del popolo birmano e per indurre il regime di Yangon ad avviare finalmente un dialogo con l'opposizione democratica. L'Italia ha attivamente sostenuto la dichiarazione della Presidenza dell'Unione Europea, che ha riaffermato nei giorni scorsi a nome dell'Unione l'intenzione di continuare ad esercitare ogni possibile pressione sul regime di Myanmar, in stretto coordinamento tra i *partners* europei. ad esempio, un *action paper* che dovrà contenere l'inasprimento delle sanzioni nei confronti della Birmania. proprio questa mattina il Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea, composto dagli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione a Bruxelles, su indicazione delle rispettive capitali, ha sottolineato l'esigenza di rafforzare il sistema sanzionatorio attualmente in vigore nei confronti del Myanmar.

ad attenersi alle esortazioni provenienti dall'Unione, nonché un appello a Cina, India ed ASEAN affinché cessino di sostenere Yangon ed esercitino sulla giunta birmana un'influenza moderatrice. Sono di queste ore, inoltre, gli ulteriori sviluppi in sede ONU: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato convocato in una riunione straordinaria ieri pomeriggio, 26 settembre, a New York, per permettere all'inviato speciale del segretario generale per Myanmar Gambari di riferire al Consiglio sugli ultimi sviluppi, prima della sua prevista partenza alla volta di Yangon su richiesta del segretario generale Ban Ki-Moon. Al termine di quella riunione, la Presidenza di turno francese ha reso, a nome del Consiglio di Sicurezza, una dichiarazione con cui ha espresso viva preoccupazione per gli ultimi sviluppi, invocato una ripresa del dialogo politico, chiesto alle autorità birmane di dar prova di moderazione ed espresso pieno sostegno ai buoni uffici del Segretario generale e del suo inviato Gambari. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno inoltre concordato, nella giornata di ieri, una dichiarazione congiunta, in cui si chiede un'immediata un'immediata iniziativa all'ONU e al Consiglio di Sicurezza, con il superamento di quelle resistenze che impedirono, nel febbraio scorso, l'adozione di un progetto di risoluzione su Myanmar. Questa è, signori senatori, l'informativa che il Governo ha ritenuto di svolgere in quest'Aula. La situazione è in costante evoluzione: notizie di agenzia indicano che, proprio in questi momenti o in queste ore, i militari hanno aperto il fuoco con armi automatiche contro i manifestanti a Rangoon. È, quindi, una situazione drammatica e preoccupante e, da quello che appare, in continua e, purtroppo, drammatica evoluzione. L'intenzione del Governo è di seguire con la massima attenzione questi sviluppi, adottando tutte le iniziative di cui vi ho già detto e le ulteriori che saranno necessarie, anche in relazione all'evolversi della situazione,

Il Governo non mancherà, naturalmente, di tenere costantemente aggiornato il Parlamento sugli sviluppi sul terreno e sui negoziati in corso nelle diverse istanze internazionali.

Presidente, colleghi, gli avvenimenti di Birmania ormai hanno avuto un impatto cruciale nelle ultime settimane, captando l'attenzione dei due colossi vicini, Cina e India, e si affacciano adesso sulla scena mondiale. La posta in gioco è altissima per la Cina, che in Birmania conta interessi economici strategici, ma è appetibile anche per l'India, che vanta legami naturali, storici e culturali con la vicina Myanmar, e ha dato il suo appoggio alla Giunta militare, per evitare un'eventuale invasione cinese. Il tutto con l'effetto assurdo di trascurare totalmente vitali diritti umani, che in questo modo rischiano grosso e, in questo contesto di giochi politici, la ribellione di tanti. Ma la protesta in atto, nata per reagire ai soprusi che il regime militare, da oltre cinquant'anni, perpetra a danno delle popolazioni, come sempre, è sfociata in atti repressivi del regime, a danno di uomini e, soprattutto, contro donne e bambini, scesi nelle piazze, accanto ai monaci buddisti, sfidando le raffiche dei colpi di arma da fuoco e i gas lacrimogeni della giunta militare. È un terribile paradosso prendere atto di simili comportamenti violenti, in un mondo che lotta per portare avanti ideali di tolleranza, libertà e democrazia. È inconcepibile comprendere simili massacri nel mondo delle

e che si basa sull'uso massiccio del lavoro forzato, sulle deportazioni di massa e finanche sull'uso di bambini soldato. Questo *status* non può essere approvato da comunità civili e democratiche, perciò sia il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che altre potenze mondiali devono intervenire per correre ai ripari. Tanto meno quest'Assemblea può esimersi dal prendere posizioni e rendersi indifferente, trascurando di aver preso all'unanimità - proprio nei giorni in cui montava la protesta in Birmania - la decisione su una mozione che impegna il nostro Governo ad operarsi in tutte le sedi internazionali per il ripristino dei diritti fondamentali dell'uomo. Vorrei ribadire che una popolazione non può subire continue prepotenze non si deve credere che la protesta sia riservata esclusivamente agli ordini religiosi, che per primi hanno messo in atto tale protesta... L'Italia deve quindi adoperarsi in tutte le sedi e presso tutti i Paesi affinché ci sia una forte pressione internazionale contro il regime di Myanmar. Del resto fanno ben sperare le ultime dichiarazioni provenienti dalla Farnesina, che sottolineano un'intesa raggiunta tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti con una dichiarazione congiunta di una immediata iniziativa all'ONU e al Consiglio di Sicurezza. Un forte appello, dunque, alle comunità

che peraltro confermano che ci troviamo di fronte ad un regime corrotto e brutale, che agisce con grande spietatezza e che non solo soffoca i diritti più elementari della popolazione ma affama anche la popolazione, come anche i dati economici che sono stati riferiti confermano. Non c'è dubbio che l'Italia debba intervenire attivamente per frenare la repressione e avviare un processo democratico. Credo che però, per poterlo fare, in qualche modo occorrerà condizionare la giunta militare, colpirne gli interessi e soprattutto provare a fermare il rifornimento di armi, compiendo tutte le pressioni politiche necessarie. È evidente che in ballo ci sono la Cina, l'India e la Russia in primo luogo, che sono i principali *partners* commerciali del Governo di Myanmar e che

molto forte, di pressione, per bloccare il sostegno che il Governo birmano ha da queste potenze. Allo stesso tempo, però, ricordo che anche i Paesi occidentali e l'Europa hanno investimenti molti forti in quel Paese, che possono quindi incidere

di persone che manifestano con il più radicale degli atteggiamenti pacifici non ci possa essere reazione adeguata oltre all'orrore e allo sdegno che ci unisce.

i passi che sta intraprendendo e di cui ci ha parlato. Sottolineo che quando, pochi giorni fa, abbiamo approvato una mozione, firmata da senatori di entrambe le coalizioni, c'era stata da parte del Governo una richiesta di attutirne il dispositivo. L'urgenza dei fatti dimostra che aveva ragione aveva ragione l'Aula a chiedere azioni incisive. Mi pare che i passi interpresi attraverso l'Unione Europea vadano verso questa direzione. Tuttavia, dobbiamo anche pensare a misure che siano efficaci. Sappiamo molto bene chi è il primo *partner* commerciale della Birmania, la vicina Cina; sappiamo molto bene che è la stessa Cina che ha impedito, sta impedendo e certamente tenterà di impedire, forse impedirà, che le Nazioni Unite prendano delle decisioni veramente forti nei confronti della Birmania. Allora, schierarsi a favore di sanzioni nei confronti della Birmania, ma contemporaneamente ignorare che violazioni dei diritti umani, forse non così spettacolari ma certamente molto più diffuse, avvengono ogni giorno in Cina, apprestarsi a celebrare con grande fasto le Olimpiadi che fra dieci mesi e mezzo metteranno la Cina e il suo regime sotto una luce certamente positiva, che ci ricorda o almeno mi ricorda quanto avvenne a Berlino nel 1936, fare questa azione sulla Birmania e non aver

di sospendere l'embargo per quanto riguarda le armi nei confronti di quel Paese, facciamo veramente un lavoro inutile: è come tentare di svuotare un contenitore d'acqua che

questo elemento minimo di civiltà che consiste nel non reprimere con le armi chi manifesta in modo del tutto pacifico, dobbiamo essere conseguenti e pensare davvero ad azioni incisive - che non vogliono dire un semplice semplice fervorino di qualche minuto davanti a qualche dirigente cinese - anche nei confronti del regime che è la causa del sostegno e della permanenza al potere della giunta birmana. In un messaggio,

i nostri corpi, ma i nostri spiriti restano intatti». Bene, noi che abbiamo i nostri corpi ben al sicuro, se non faremo qualcosa di veramente incisivo, difficilmente manterremo i nostri spiriti intatti.

la situazione è veramente tragica

Abbiamo ascoltato che i militari hanno aperto il fuoco contro i monaci e contro i dimostranti,

Ricordiamo che il premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, figlia del padre della patria birmana Aung San, vive agli arresti domiciliari. Non vi è dubbio che la comunità internazionale

per motivi di carattere economico e strategico, in qualche modo sostengono il regime, direttamente o indirettamente.

Signor Presidente, signor Vice ministro, stiamo seguendo con apprensione e preoccupazione gli sviluppi della situazione nel Paese asiatico e, a nome di tutto il Gruppo Per le Autonomie, intendo esprimere la nostra solidarietà al popolo, ai monaci birmani, che da settimane protestano in modo pacifico contro la giunta militare del potere nel nuovo Myanmar o ex Birmania. Non intendo soltanto esprimere pieno sostegno a quel popolo, ma anche ringraziarlo per l'esempio di coraggio civile che offre al mondo con la sua protesta non violenta. Come denunciato dalla Croce Rossa e da altre organizzazioni internazionali e come appena confermato dal Governo, per voce del vice ministro Danieli, il regime militare contro cui manifestano da settimane costituisce uno dei casi peggiori di regime in cui siano violati diritti umani fondamentali. Esprimiamo la nostra forte preoccupazione per questo brutale regime nella ex Birmania e quel che più ci preoccupa ora è il dover apprendere che le autorità militari hanno dato seguito alla loro minaccia che da ieri cerca di reprimere con la forza queste pacifiche manifestazioni. Oltre ai feriti, si registrano già dei morti e molti arresti di monaci. A nome del Gruppo Per le Autonomie, ringrazio pertanto il Governo e il vice ministro Danieli che si è subito attivato e lo sosteniamo e lo sosteniamo nello svolgere una immediata azione sugli organismi internazionali per accentuare l'isolamento del regime militare birmano e fermare subito questo ricorso alla forza. Supportiamo il Governo anche nell'impegno direttamente rivolto alle sedi europee e nel sostegno politico e materiale nei confronti delle organizzazioni democratiche sindacali e politiche della ex Birmania, oggi dichiarate fuorilegge. importante, come già sottolineato da vari oratori, sensibilizzare i Governi di India e Cina, principali *partner* commerciali della Birmania, affinché favoriscano una soluzione pacifica della protesta ed una reale democratizzazione del Paese. Chiediamo inoltre di esercitare pressioni affinché vengano liberati il più presto possibile tutti i prigionieri politici, compreso il premio Nobel della pace Aung San Suu Kyi.

del popolo birmano e sostengono questa lotta non violenta per la libertà nel loro Paese. Ringraziamo il Governo e il vice ministro Danieli per il suo operato il suo operato e ci auguriamo che si arrivi ad una soluzione (anche se le notizie appena date in diretta dal vice ministro sono molto preoccupanti), che sia evitato il bagno di sangue e che la giunta militare cessi il controllo del Paese. Approfitto dei cinque minuti a mia disposizione per portare all'attenzione del Governo e dell'Aula una denuncia fatta da un gruppo di associazioni internazionali per i diritti, tra le quali *Amnesty International* e *Saferworld*, in riferimento ad un armamento che l'India si apprestava e si appresta a dare alla Birmania, che contiene - nonostante l'embargo dell'Unione Europea sugli armamenti in relazione alla Birmania - atti e atti e costruzioni di sei Paesi europei, tra cui anche l'Italia da parte dell'azienda elettronica Aster. Dico subito che questi prodotti non sono venduti alla Birmania, ma sono dati all'India per un nuovo elicottero d'attacco, un elicottero prodotto in India, ma che non potrebbe funzionare senza questi componenti essenziali provenienti dai Paesi europei, in particolare Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Svezia. Questo potrebbe invalidare, anzi invalida l'embargo che nel 1988 l'Unione Europea ha correttamente stabilito sulla Birmania in relazione agli armamenti, proprio per le gravissime violazioni

affinché il controllo, specialmente sulle triangolazioni in riferimento agli armamenti, venga effettuato con maggiore attenzione, perché se è vero - ad esempio l'azienda italiana credo che faccia solo freni

Quindi, vi è il rischio che comunque, anche indirettamente, nonostante la volontà politica dell'embargo dichiarato, arrivino armi agli oppressori del popolo birmano, come - devo dire - arrivano armi comunque e, sempre con la triangolazione, ovunque nonostante gli embarghi. Questo caso vale anche per gli Stati Uniti che pure hanno stabilito l'embargo, ma non hanno messo la clausola all'India - perché in questo caso si parla dell'India - del divieto di vendita alla Birmania del materiale bellico dato all'India.

Credo che sia da valutare con molta attenzione la proposta degli organismi internazionali affinché una missione del Consiglio di sicurezza dell'ONU - come già ci ha anticipato il Vice ministro - sia inviata, ma con una determinazione forte, per far capire che non sarà tollerato un altro bagno di sangue, come successe, con 3.000 morti, anni fa. Purtroppo le notizie che ci ha portato il Vice ministro vanno in un'altra direzione,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da mezzo secolo uno dei Paesi più ricchi dell'Asia, la Birmania, fornitore di petrolio, gas, giada e rubini, teak e legnami pregiati, è oppresso da una dittatura sanguinaria. A distanza di quasi vent'anni dalla repressione cruenta operata dagli squadristi dei generali della Giunta militare al potere ai danni degli studenti, delle minoranze etniche, degli insorti delle foreste orientali, è ritornata prepotente la richiesta, l'urlo di libertà e democrazia, questa volta invocato dai monaci che sono scesi in piazza a Yangon, lasciando il tempio di Shwedagon e invadendo pacificamente la città. La protesta di questi giorni non è solo una rivendicazione di miglioramenti economici; certo le richieste di migliori condizioni di vita, tese ad avere i benefici di ciò che il Paese produce, sono la benzina che alimenta le manifestazioni di piazza. Vedere questa enorme massa di risorse finire sfruttata a beneficio dei due grandi protettori della Giunta militare birmana, che sono la Cina e l'India, è per i birmani sempre più insopportabile. La protesta - come abbiano detto - è la richiesta di veder soddisfatto il primo, unico valore inalienabile per ciascun uomo: la libertà. Purtroppo i fatti di ieri hanno ripetuto il copione del 1988, con almeno cinque morti (qualcuno riporta sei), di cui uno è un monaco, decine di feriti e trenta arresti. I militari stanno tentando di stroncare sul nascere questa ennesima richiesta di libertà. Hanno cominciato con il deportare San Suu Kyi, il premio Nobel per la pace, sfilandola anche fisicamente dall'immagine della protesta. La repressione violenta è per il regime militare la strada sulla quale intende bloccare ogni cambiamento in favore della conquista degli elementari diritti umani delle popolazioni birmane. Oggi, dopo dieci giorni di manifestazioni continue, con decine di migliaia di monaci nelle piazze e centinaia di migliaia di cittadini al loro seguito, la situazione sembra volgere verso la soluzione più nefasta. Il regime tiranneggia da decenni il Paese, costringendo i dissidenti politici ai lavori forzati o rinchiudendoli in gabbie per cani nella prigione di Insein. I reati di pensiero in Birmania sono puniti con dieci anni di carcere ed è considerato tale semplicemente scrivere una lettera con contenuto non autorizzato o volantineggiare e fare opera di proselitismo. Il regime si regge sulla politica del terrore e dell'esclusione politica. Da anni le popolazioni sono costrette a fuggire dai villaggi, dove l'esercito brucia le case e uccide chi tenta di farvi ritorno. Il Governo è fatto pressoché di generali. In questo quadro, le democrazie occidentali si sono mobilitate non violenta per la promozione dei diritti umani e la democrazia, rivendicate da un popolo che è sceso in piazza per chiedere libertà e democrazia, sia sostenuta dall'intera comunità internazionale e si arrivi presto alle elezioni, quelle elezioni che la Lega nazionale per la democrazia vinse quasi vent'anni fa, conquistando 392 seggi su 485. A capo di quel movimento vi era il premio Nobel per la pace San Suu Kyi, che oggi è sottratta coercitivamente persino dalla protesta e tradotta in carcere. Il Presidente degli Stati Uniti, fedele al suo "*The liberty speech*", discorso della libertà, di pieno sostegno alla crescita dei movimenti democratici in ogni nazione e in ogni cultura, con l'obiettivo di porre fine alla tirannia nel mondo, ha dal pulpito dell'ONU lanciato un ammonimento e annunciato l'inasprimento delle sanzioni contro il regime birmano e chi lo sostiene e un bando sui visti dei responsabili delle violazioni più plateali dei diritti umani. Il presidente francese Sarkozy ha platealmente ricevuto all'Eliseo Sei Win, il *leader* dell'Unione birmana, quel politico che nel 1989, dopo aver vinto le elezioni, fu cacciato in esilio dai militari, sottolineando in questo modo che Parigi parla solo con chi è stato legittimato dall'investitura popolare, chiudendo la porta in faccia ai tiranni di Yangon. Gordon Brown ha scritto anche al Presidente portoghese della UE chiedendo che l'Europa inasprisca le sanzioni economiche alla Birmania. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale auspica che la situazione birmana possa evolversi positivamente arrivando alle libere elezioni, senza ulteriori bagni di sangue. Purtroppo, il volto duro dei generali del Myanmar, che hanno imposto il coprifuoco dalle ore 9 di sera alle ore 5 di mattina, insensibili agli appelli della comunità internazionale che chiede equilibrio, moderazione e dialogo, non lascia ben sperare. Il silenzio, per non dire l'ostilità, di Cina e India manifestatosi anche questa notte nella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è l'espressione cinica di queste due superpotenze, che antepongono i loro interessi loro alle legittime richieste del popolo birmano. Il Consiglio di Sicurezza non ha trovato un'intesa sulle misure più efficaci e le sanzioni contro la Birmania. In particolare, Russia e Cina si sono opposte alle sanzioni. Questa notte il loro no, unito a quello dell'Indonesia, ha impedito al Consiglio di raggiungere un accordo. India, Cina e Russia preferiscono la stretta alleanza al regime del Myanmar per continuare nel loro progetto di colonizzazione di quel Paese, nel quale hanno investito in modo ingente per sfruttarne le materie prime. Esse sarebbero le uniche Nazioni in grado di disarmare la giunta militare, ma si sottraggono a questa responsabilità, preferendo tutelare il loro strategico alleato anche se da una parte continua ad essere un regime sanguinario e sempre più repressivo. Signor Presidente, Alleanza Nazionale prende atto dei provvedimenti assunti dal Governo unitamente ai Governi della comunità internazionale, e in particolare dell'Europa, atti ad indurre la giunta militare a non perseverare nella violenta repressione in atto. Invitiamo altresì il Governo a prendere direttamente tutte le azioni, compreso l'embargo, atte a costringere la Birmania ad un cambio di regime, imboccando finalmente la strada della democrazia, della giustizia e della pace. *(Applausi dal

Anch'io, a nome del Gruppo Sinistra Democratica, ringrazio il Governo e il vice ministro Danieli per la sollecitudine con la quale è venuto a riferire in Aula e per le iniziative esposte, peraltro già avviate dal nostro Governo nei confronti

tragedia che potrebbe avvenire. Dobbiamo evitare il 1988, anche se le notizie adesso date dal Vice ministro sono drammatiche; se non ho capito male, è stato addirittura ucciso un fotografo giapponese,

Dobbiamo evitare che questa rivolta rimanga un urlo nel silenzio, come lei ha detto ed io voglio ripeterlo: questo silenzio assordante della politica internazionale che quando ha parlato di ingerenza umanitaria ha sempre rivolto lo sguardo da un'altra parte quando si trattava di Birmania.

e quindi, da questo punto di vista, penso che occorra continuare e passare ad un'altra fase. Servono sanzioni vere, non simboliche come quelle sui visti preannunciate dallo stesso presidente Bush, che ha tuonato molto ma ha prodotto poco.

della Birmania da parte di questi importanti attori a livello internazionale, tanto più nella propria regione. La forza del Governo di Yangon, comunque, è consistita in questi anni anche nel rastrellamento di tanti e grandi investimenti stranieri, stranieri, come quello della Total, della Fina, dell'Unocal, che hanno investito 2 miliardi di dollari nello sfruttamento del gas naturale di quel Paese. Quando si investono 2 miliardi di dollari a volte si rischia di chiudere gli occhi sulla repressione e sul lavoro forzato imposto,

un'altra piazza insanguinata, quella della ex Birmania. Viviamo nel paradosso: sangue chiama sangue. L'altro giorno nove morti ammazzati e altri due, quasi ammazzati, in Afghanistan. Sei monaci buddisti ieri uccisi a Rangoon, l'ex capitale birmana, assieme, dicono le agenzie, a decine e decine di cittadini sotto il fuoco della polizia aperto ad altezza d'uomo. Cosa diciamo rispetto al vile ed efferato episodio di cui ci occupiamo? Diciamo che siamo di fronte ad un caso di atrocità? Ripetiamo la solita solidarietà alle famiglie e al popolo dei sei buddisti assassinati? Ci esibiamo, facendo a gara nelle auliche espressioni di cordoglio e di buoni propositi? No, vediamo finalmente di uscire dall'ovvio e dalla solita, ripetuta declamazione. Diciamo, chiaro e forte, una sola cosa: nessuno, proprio nessuno, può pensare che la questione dell'ex Birmania sia di quelle per cui occorrerà far parlare prima o poi, ancora una volta, le armi, quelle della NATO ovviamente, sotto l'egida e l'assenso dell'ONU. Noi nutriamo terrore verso la giunta militare birmana, solida nella sua efferatezza, consolidata nei suoi circa 45 anni di dittatura. Nutriamo sgomento ancora oggi per le 3.000 persone ammazzate nel 1988 dal pugno di ferro birmano contro le manifestazioni di uomini e donne inermi a favore della democrazia di quel Paese. Noi sentiamo inquietudine e sorpresa per lo spostamento della capitale birmana a 240 chilometri a Nord di Rangoon, che venti non bloccati da barriere ci indicano che questo potrebbe essere tradotto in un ammassamento di truppe al sud del Paese, in vista di una repressione a tappeto di monaci e di popolazione in rivolta. Di fronte a tanta cupa prospettiva, tutti assieme facciamo nostro l'invito rivolto da Bush all'ONU di tornare alle Nazioni Unite, ai suoi princìpi fondanti e al centro delle discordie - ovunque essi siano, però, ecco il punto - nel senso dell'esercizio da parte dell'ONU della massima moderazione e del metodo del dialogo con tutte le parti, nell'unica prospettiva di tentare di dar vita, di ridar vita, ovunque e sempre quindi, anche in ex Birmania, ad un metodo che realizza un costante e duraturo processo di riconciliazione all'interno dei popoli e tra i diversi popoli. Conclusione, Presidente: l'occasione che ci occupa credo la spenderemo bene noi di questa Assemblea se nel cuore e nella mente di ciascuno di noi facciamo prevalere sulle facili suggestioni dell'uso delle armi, per il superamento delle discordie, la ragionevole e civile moderazione della diplomazia e delle relazioni internazionali. Nel solco di tale prospettiva osiamo introdurre l'invito al Governo di volersi dedicare, con la partecipazione ed il concorso del Parlamento, alla rimeditazione sui nostri impegni militari nelle varie regioni del mondo, al fine di stabilire se il nostro Paese debba e possa continuare ad essere coprotagonista in armi in aree del mondo, sempre più numerose e per periodi di tempo sempre più estesi, tendenti a superare la durata dei conflitti mondiali e regionali dell'ultimo secolo.

Presidente, onorevoli colleghi, siamo oggi qui riuniti per discutere dei fatti che stanno in queste ore insanguinando

la posizione politica del Gruppo UDC al Senato della Repubblica, non solo per manifestare una forte preoccupazione - che mi sembra comune a tutti i Gruppi parlamentari ed ai colleghi che sono intervenuti

scarsa attenzione di Paesi come l'Italia, che hanno problemi a sostenere nei fori internazionali una politica estera credibile, nel tentativo di contenere la propria maggioranza all'interno del Paese. Proprio per questo abbiamo difficoltà, ma ciò non impedisce al nostro Gruppo di sostenere l'azione del Governo

nei confronti della Cina e dell'India, perché ritengo che questi due Paesi, oltre che la Russia, possono svolgere un ruolo molto importante per sedare questa protesta e per consentire, non solo ai monaci ma a tutti i civili che si stanno battendo per i diritti umani, di poter avere dei cenni di riscontro. Devo sottolineare anche l'importanza, in questo caso, di Internet e dei *blog*, che hanno consentito alla comunità internazionale di conoscere

fare un appello affinché il Governo di Pechino possa esprimere una sua posizione più forte, meno generica di quanto avvenuto fino ad ora.

Governo, dall'Europa, dai fori internazionali, dalle Nazioni Unite. Dobbiamo ottenere tre importanti risultati, caro vice ministro Danieli:

che affama quella gente, che sta battendosi non solo per la sua libertà ma anche per la libertà di quel popolo e delle future generazioni.

della italianità e della diplomazia italiana. Non siamo un superpotenza militare, siamo una superpotenza culturale e diplomatica, quindi la nostra azione può essere quella di avvicinare con la nostra mediazione Paesi come la Cina, l'India e la Russia, affinché anche con un'azione bilaterale l'Italia possa raggiungere questi obiettivi.

se c'è una cosa che ci insegnano queste giornate drammatiche a Rangoon e in tutta la Birmania è che quanto previsto nel libro che pubblicò anni fa Aung San Sun Kyi, "Liberi dalla paura", forse oggi, in un certo senso, si sta materializzando. questo popolo vive sotto un regime spietato, abbiamo già avuto occasione di parlarne la scorsa settimana e anche oggi in questa Aula, però qualcosa di nuovo sta accadendo. È un popolo che forse, grazie alla forza spirituale di centinaia di migliaia di monaci e monache buddiste che rappresentano l'ossatura e la continuità della storia di quel Paese, ha ripreso il coraggio di scendere in piazza, di chiedere finalmente una transizione verso la democrazia, nel rispetto delle libertà e dei diritti umani; lo fa con metodi non violenti, quelli propri della filosofia e della religione buddista e sarebbe una grande sconfitta per tutti noi, che crediamo nella non violenza come pratica quotidiana, anche nella politica, se questa volta non si riuscisse a dargli voce rappresentanza e forza per continuare nella sua opera, che oggi sembra impossibile e improba.

Siamo molto confortati dalle parole del vice ministro Danieli dalle quali emerge che finalmente il Governo ha compreso di aver compiuto un grave errore ad invitare dei funzionari birmani ad un corso di formazione sui diritti umani. è stato commesso un errore di valutazione la scorsa settimana quando ci è stato chiesto di ammorbidire una mozione parlamentare che, purtroppo, forse anticipava quello che oggi andrà fatto. fatto. Se il Governo avesse dato seguito alle nostre richieste probabilmente oggi avrebbe avuto maggiore forza politica nel chiedere quello che sta chiedendo. Ma oggi non è il momento di analizzare tali questioni. Mi unisco alla richiesta avanzata da molti in quest'Aula di escogitare, di pensare anche ad altri strumenti per esercitare maggiore pressione non solo sulla Birmania, ma anche sui Paesi che oggi la proteggono politicamente, quei Paesi che ieri al Consiglio di Sicurezza hanno usato il pretesto inaccettabile del diritto di non ingerenza, quando poi in effetti interferiscono - eccome - nella vita politica, economica e sociale di quel Paese! A tal riguardo, si ricordi che la Cina oggi ha una cosa a cuore: i giochi olimpici ed ha a cuore la sua reputazione a livello internazionale. E l'India ha un'altra cosa a cuore: il fatto di diventare un *partner* strategico anche dell'Italia, dal punto di vista industriale, commerciale ed economico. Come ha affermato il senatore Silvestri, oggi indirettamente

fare le debite considerazioni anche per quanto riguarda le sanzioni economiche e commerciali. Vorrei ricordare peraltro che l'Italia continua ad importare prodotti naturali ed altre merci dalla Birmania.

forse sarà il caso che l'Europa faccia la sua parte dando seguito alle raccomandazioni contenute in una risoluzione d'urgenza del Parlamento Europeo di due settimane or sono che oggi mi sembrano recepite *in toto* anche dal Governo italiano, cosa di cui assolutamente

da tutte le senatrici che oggi in questo Senato manifestano con un documento firmato da tutte la loro solidarietà ad Aung San Suu Kyi e alle monache buddiste. Mi sembra anche questo un elemento molto importante che speriamo possa aggiungere forza alla forza che il popolo birmano oggi sta dimostrando a tutto il mondo.

Due settimane fa in quest'Aula per iniziativa di 74 senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari il Senato della Repubblica approvava all'unanimità una mozione per la liberazione di Aung San Suu Kyi e il rispetto dei diritti umani in Birmania. Di lì a poco migliaia di monaci, monache e studenti, il popolo birmano, hanno scosso il mondo manifestando per la libertà della Nazione e la stessa Aung San Suu Kyi si è unita alle loro preghiere. Così lontani nello spazio, così vicini nella coscienza civile comune. Oggi siamo qui con l'animo in angoscia per la violenta repressione in atto, gli spari sulla folla, le uccisioni, l'arresto dei monaci e degli oppositori del regime, la caccia anche agli occidentali negli hotel, mentre incerta è la sorte di Aung San Suu Kyi, *leader* della Lega per la democrazia, premio Nobel per la pace. ha anche notizia di militari che si sono rifiutati di aggredire i monaci. Signor Presidente, signor Vice ministro, nel dialogo che qui si svolge tra la volontà del Parlamento e le intenzioni e le scelte del Governo è racchiusa tutta intera la volontà dell'Italia e del nostro popolo in questo momento. Sia liberata Aung San Suu Kyi, sia fermata subito la repressione, si apra il dialogo di riconciliazione nazionale sotto l'egida delle Nazioni unite, l'inviato speciale Gambari entri subito a Rangoon. L'impegno del nostro Governo deve essere determinato e tempestivo. Mentre noi siamo qui, i monaci, anche giovanissimi, sono picchiati e arrestati, un'intera generazione birmana è di nuovo a rischio dopo il massacro del 1988, il popolo è stremato dalla paura e dalla povertà. Il Presidente del Consiglio ieri ha dichiarato il fermissimo impegno del Governo, ribadito dal Ministro degli esteri e oggi qui dal Vice ministro. Vi sono momenti nella storia in cui siamo coinvolti nei cambiamenti con tutto ciò che siamo, i nostri valori, le nostre responsabilità, noi viviamo uno di questi momenti, perché mai nella storia dell'umanità le sorti della democrazia e dei diritti umani sono stati così globali, senza confini, interpellando la coscienza di tutti nel mondo. Oggi siamo tutti birmani, oggi più che mai sentiamo l'urgenza delle Nazioni Unite e del loro ruolo, è necessario che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si muova con tutto il suo potere, superando ancora i freni e i veti, rivelatisi anche nelle ultime ore. L'Unione Europea (il Parlamento è già andato in questa direzione con voto unanime in queste ore) rafforzi le sanzioni economiche e commerciali nei confronti del Myanmar, senza eccezioni, ma insieme con queste la sanzione deve essere soprattutto politica, il nostro Governo si adoperi in tutte le sedi e rappresenti alla Giunta del Myanmar la volontà dell'Italia, chieda alla Giunta di liberare i monaci e i democratici arrestati: dove sono? Il mondo intero guarda e chiede conto. In secondo luogo chiediamo a lei, signor Presidente dell'Assemblea, di adoperarsi perché una delegazione del Senato della Repubblica possa incontrare semplicemente Aung San Suu Kyi in nome del popolo italiano, ma una politica a tutto campo è indispensabile per la svolta politica in Birmania. La Cina e l'India, oltre alla Russia, come si vede in queste ore, sono interlocutori fondamentali, lo abbiamo detto tutti. Io stessa qualche settimana fa in Cina con l'Associazione degli amici parlamentari della Cina ho avuto occasione, parlando con le autorità cinesi, di parlare di Aung San Suu Kyi e della Birmania e di chiedere che cosa ne pensavano, confidavo non nella risposta, ma almeno nell'ascolto. L'Unione Europea e gli Stati Uniti usino tutta la loro influenza, del resto come è avvenuto in queste ore, con una rapida posizione comune per costringere la Giunta militare a prendere atto che il corso della storia in Birmania deve cambiare dopo 45 anni di dittatura. Il mondo globale sa che non vi possono più essere il mercato disgiunto dai diritti umani fondamentali, i commerci disgiunti dalla democrazia in Asia, la democrazia in Asia e i diritti umani nascono anche dalle sorgenti millenarie della spiritualità buddista, non violenta, che oggi con la testimonianza corale dei monaci sta parlando al mondo. Forse la via dell'Asia è la democrazia, è un grande segnale per l'intera area asiatica e per il mondo. Nel 2008 vi saranno i Giochi olimpici a Pechino, simbolo stesso del dialogo e dopo nulla sarà come prima; bisogna parlare con la Cina oggi anche di questo. La Birmania oggi è la porta per il futuro dell'Asia, fondato sui valori della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani, anche noi siamo chiamati in causa nelle nostre responsabilità. Ha scritto Aung San Suu Kyi: «Il sogno di una società governata da amorevole gentilezza, razionalità e giustizia è vecchio quanto l'uomo civilizzato. Questo sogno è obbligatoriamente irrealizzabile? Io credo di no e per questo lotto con tutte le mie forze». Oggi vorremmo dire ad Aung San Suu Kyi: «Noi la pensiamo come lei, coraggio», in ogni parte del mondo la mobilitazione è grande, si moltiplicano appelli delle donne, dei capi di Stato, anche delle loro mogli, come la moglie di Bush, dell'opinione pubblica. Nessun Paese è un'isola, il destino di ogni popolo appartiene a quello dell'umanità, un destino unico di libertà. Lo sappia il popolo birmano, lo sappiano gli esuli e i profughi al di qua del confine: l'Italia è con voi; il mondo è con voi, non siete soli. Oggi, consegniamo al Governo la responsabilità di rendere concreti e immediati questo sentimento e questa volontà. Credo che, a questo punto, essendo terminato il dibattito, la Presidenza possa sottolineare, senza forzare niente, che vi sono state una fortissima condivisione del giudizio sui fatti birmani e - devo dirlo - anche una partecipazione, da parte delle senatrici e dei senatori che hanno parlato, rispetto agli sviluppi di una situazione che sta diventando drammatica.

nella dovuta considerazione. Come sapete, l'ONU, il Parlamento europeo a stragrandissima maggioranza ed il nostro Senato, con questo dibattito, stanno compiendo ogni sforzo per bloccare questo che si delinea ormai come un vero e proprio massacro e garantire, ove sia possibile - e speriamo che lo sia - attraverso tutte le forme diplomatiche e l'intervento diretto, anche del Senato della Repubblica, la liberazione di Aung San Suu Credo che il Senato abbia dimostrato una profonda partecipazione alle vicende di questo popolo con il dibattito a cui abbiamo dato corso in questa mattinata.

nella società italiana il disprezzo verso i parlamentari. È davvero molto grande: si tratta di un fenomeno che, a mio giudizio, dovrebbe preoccuparci che esso, purtroppo, è stato alimentato da errori e inadempienze di cui certamente siamo responsabili, ma so anche che, in questo momento, si rivolge a molte persone che non lo meritano.

svuotata. Signor Presidente, ritengo che i colleghi non si rendano conto di cosa questi episodi significhino nel confermare quello stato di disprezzo nei nostri confronti che sta crescendo nel Paese, cosa di cui profondamente mi dolgo. *(Applausi dei

Grazie,